finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato,

per così dire stagionale con cui il Senato sta affrontando un disegno di legge come questo, su una riforma di grande rilievo, come quella dell'ordinamento forense, non dipende né da una distrazione della Presidenza del Senato né da cattiva volontà di questa Assemblea, ma dal grave errore originario di impostazione di questo provvedimento. Due anni fa, nel novembre 2008, il ministro Alfano, al Congresso nazionale forense di Bologna, ha fatto agli avvocati un discorso che suonava sostanzialmente se voi mi portate un disegno di riforma sul quale concordino tutte le componenti e le voci dell'avvocatura, io mi impegno a farlo passare in Parlamento. Con questo discorso il Ministro mostrava di non tenere nel minimo conto il fatto che - dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo, nel quale l'Ordine degli avvocati era al tempo al tempo stesso ente pubblico e organo unico di rappresentanza degli interessi economici e professionali degli avvocati la disciplina della professione forense non è più posta dallo Stato nell'interesse prioritario degli avvocati, bensì è posta principalmente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e della collettività. Sulle linee e sui contenuti della riforma, dunque, non poteva certo bastare un accordo limitato alle componenti interne dell'avvocatura. In realtà, quell'accordo in seno al ceto forense che il ministro Alfano richiedeva non è stato affatto raggiunto: ad esempio, non sono affatto d'accordo con questo disegno di riforma i giovani avvocati.

delle imprese, l'Antitrust e l'interesse ad un corretto svolgimento della concorrenza nel mercato dei servizi forensi e legali. Di tale interesse, che avrebbe dovuto costituire il punto di riferimento principale per questa iniziativa legislativa, il ministro Alfano si è invece totalmente dimenticato, con il risultato che, appena partito, il disegno di legge si è incagliato. Così stando le cose, chiedo al Governo di chiarirci se, nei cinque mesi che sono trascorsi dall'ultima volta in cui ci siamo occupati di questo provvedimento, sia maturata un'impostazione più meditata, una considerazione più attenta degli interessi che questa nuova legge dovrà proteggere. Vorrei che ci venisse anche chiarito quali modifiche ne derivano, secondo gli intendimenti del Governo, nelle linee portanti del disegno di legge.

a che siano inserite le seguenti parole: «I costi per le attività previste sono posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di formazione».

esplicitava che non vi fossero oneri a carico dello Stato, ma certamente non che i suddetti oneri dovessero essere a carico dei partecipanti ai corsi. Poiché i consigli dell'ordine, i CNF, hanno una loro caratterizzazione economica certamente autonoma rispetto allo Stato, credo che questi organismi di categoria, peraltro istituzionali, possano tranquillamente assumersi gli oneri

non appare potersi svolgere in maniera gratuita, è chiaro che qualcuno le risorse per svolgerla dovrà tirarle fuori. Siccome stiamo parlando di organismi che appartengono all'area rientrano tra gli enti pubblici, qualsiasi onere, più o meno determinante nello svolgimento del corso, comunque trae origine da risorse pubbliche.

questo è pacifico. Allora, noi dobbiamo votare l'emendamento 10.200 che non ha nulla a che fare con quanto detto dal collega Fleres. Quando ci arriveremo, parleremo dell'altro

e, quindi, per coloro che vogliono partecipare ad attività di formazione. Esiste poi una serie di corsi, pubblicizzati anche su Internet, a carattere gratuito. Io non riesco a comprendere se stanno compiendo questa attività in violazione di norme di legge; non mi con questo emendamento venga affermato il principio che non si pongano ulteriori oneri a carico dello Stato. Se i consigli dell'ordine si finanziano in parte

su un articolato di 66 articoli. Quindi, abbiamo approvato un articolo su 11. Di questo passo, facendo una previsione esoterica, occorreranno 2.000 giorni per completare l'esame di questo provvedimento di legge, ovverosia sei anni. Ebbene, alcuni colleghi più competenti di me mi dicono che questa legislatura non è destinata a durare tanto e che forse durerà meno di sei anni. Allora io mi domando se questo sia l'ulteriore giorno nel quale il provvedimento viene portato qui come tappabuchi, perché questo Senato non ha

è uscito malformato dalla Commissione e ci viene qui sottoposto nell'incertezza totale, sia della maggioranza che dell'opposizione. Noi non vogliamo essere ulteriormente presi in giro! una dignità di questo Senato il sostegno di 15 senatori

la questione, che all'apparenza potrebbe sembrare di un dettaglio linguistico, è invece questione che attiene a temi di carattere generale sulla natura della professione forense e sulla natura stessa della amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Riepilogo in poche parole il contenuto dell'emendamento e dirò qualcosa sul suo significato. La norma di cui al disegno di legge che discutiamo recita che «L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti». chiede che si aggiunga un ulteriore elemento, a nostro modo di vedere fortemente qualificante di una rilettura della natura della professione legale nel quadro del nostro sistema. Tale aggiunta è: «e dell'amministrazione della giustizia». L'aggiunta in questione suscita, o può suscitare - ne siamo perfettamente consapevoli - obiezioni, a prima vista, in apparenza, anche fondate, su un'eventuale intenzione di attribuire un contenuto etico o eticheggiante alla professione forense, e il mio intervento è appunto finalizzato a sgombrare il campo da questo tipo di preoccupazioni. Risparmio naturalmente a lei, Presidente, e all'Assemblea un *excursus* storico sulla natura e sulle funzioni della professione legale; tuttavia, ci preme sottolineare

collocata in un quadro di garanzie ordinamentali, e la funzione del singolo avvocato nel momento in cui egli esercita la sua funzione e cioè difende il cliente. Non v'è alcun dubbio che nell'esercizio della professione e del singolo procedimento, nell'esercizio della singola difesa, il fondamentale criterio, diremmo la stella polare, per l'esercizio della professione debba essere e non possa essere altro che l'interesse del cliente. La questione però è quando si passa dalla valutazione del comportamento deontologicamente rilevante del singolo, finalizzato - ripeto -soprattutto alla difesa del singolo cliente,

sistemico, l'amministrazione della giustizia, che non è il criterio di ispirazione della condotta del singolo avvocato ma deve essere - vi ricordo che parliamo

poi la facondia ha preso la mano e abbiamo ascoltato molto volentieri un'elaborata e dotta costruzione delle sue ragioni. Cambio pertanto il parere precedente

in qualche modo abbiano legato, ingabbiato, bloccato e - come dice il sottotitolo - soffocato l'economia italiana: «Se con 230.000 iscritti all'albo forense importiamo consulenza legale, se non esiste la meritocrazia, se la burocrazia è pletorica e inefficiente, se la culla del diritto ne è diventata la bara, se ogni legge che entra in Parlamento ne esce finendo col dare più potere a quelli cui avrebbe voluto ridurlo, se persino il mondo dello sport è afflitto da periodiche scosse telluriche. Se, cioè, la vita italiana è costellata da tanti scandali che si ripropongono con ciclica periodicità e con ossessionante ripetitività, non può trattarsi di vicende svincolate tra loro ma deve ragionevolmente ritenersi che vi sia una radice comune, una causa non rimossa che trascende i singoli "orticelli". Per fare la storia delle professioni occorre partire proprio dagli avvocati, non solo per la primogenitura della regolamentazione alla quale si sono richiamati tutti gli ordini professionali istituiti successivamente, ma perché il mercato, per essere tale, ha bisogno del diritto. Mercato e Diritto sono "inscindibilmente legati: nascono, si sviluppano e muoiono insieme". La professione forense, quindi, per la "strategicità" "strategicità" e per la sua interferenza con la giustizia, servizio essenziale per un società che voglia dirsi civile, costituisce l'emblema, la metafora ideale per leggere le strutturali inefficienze del Paese».

Con questo disegno di legge e, in particolare, con l'articolo 10 e il suo secondo comma, che con l'emendamento 10.202 intendiamo sopprimere, si va esattamente nella direzione dirigistica di una legge che muove da un mercato

ci si rivolge all'avvocatura di altri Paesi dell'Unione europea), per continuare a mantenere questo orticello, lo ingabbia ulteriormente a tutela di chi è già dentro questo mercato, ovviamente a svantaggio di quelli che invece ne sono fuori. L'intervento è di tipo dirigista: se questa è la torta, continuate a dividerla tra di voi, e che non intervenga qualcuno di nuovo a sottrarre delle fette di torta.

chi è in grado di sapersi conquistare la propria clientela e di portare avanti la propria attività professionale deve poterlo fare.

perché incomincia a elencare una serie di figure che sono esentate. Credo che sia utile ricordare chi volete esentare dall'obbligo di formazione; soprattutto, dovrete anche rendere conto del perché

1? Si menzionano i presidenti di provincia e gli assessori provinciali. Quale formazione hanno gli assessori provinciali o i consiglieri provinciali nell'ottica dell'interesse dei loro clienti? Il fatto

Signore e signori del Senato, intervengo su questo emendamento e poi non interverrò più.

che - a mio parere - ha dimostrato in questa sede una intima contraddizione con quanto ha sostenuto più volte, ripetutamente e pervicacemente, la minoranza, la cui convinzione è che nell'Aula del Senato vi sarebbe semplicemente una mortificazione del Senato perché si passerebbe soltanto unanimemente a votare provvedimenti

con un'attenzione particolare a quanto dice ciascuno di noi rispetto ad una norma molto dettagliata ed articolata, che ha aspetti

mettere riparo a quello che ha fatto male la Commissione. Ammettiamolo pure, senatore Livi Bacci. La Commissione non ha lavorato abbastanza bene, e ce ne scusiamo - ho fatto parte del Comitato ristretto - e chiediamo a voi di correggerci, di invitarci ad una meditazione ulteriore, ad accettare o a rifiutare un emendamento. Questo per quanto riguarda la contraddizione che avevo rilevato nelle parole del senatore Livi Bacci. In ordine all'intervento della senatrice Poretti, la invito ad quando si scatena contro il comma 2 dell'articolo 10 e chiede perché devono essere esentati dalla formazione continua, per esempio, i parlamentari, le faccio presente che i parlamentari hanno una formazione continua anticipata perché, se fossero attenti, come sta attento il professor Livi Bacci, in questa sede creiamo le leggi prima ancora che siano pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. E a me sembra questo abbastanza sufficiente. Lo stesso può dirsi per i consiglieri regionali perché ci sono le legislazioni regionali. Lo stesso può dirsi per i parlamentari europei che, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, producono una serie di normative europee che stanno a noi, qualche volta, come un giogo sul collo, col massimo rispetto per l'Unione europea. Per quanto riguarda invece i sindaci delle grandi città, abbia pazienza:

10 abbiamo anticipato una misura che ieri è stata ulteriormente modificata in 1a Commissione, cioè una sorta di lodo Alfano per almeno due cariche dello Stato che non hanno bisogno di una preparazione continua ma che per l'appunto non sono esentate da questo comma 2: il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei ministri devono invece continuare a fare una preparazione quotidiana.

con rispetto parlando, di questa misura: mi pare che, ogni volta che si affronta un comma di questo sterminato articolato - lo ricordava poco fa il senatore Longo ci sarebbe bisogno di recuperare un lavoro in Commissione, visto e considerato che il prodotto finale dello sforzo avviato all'inizio di questa legislatura forse non è all'altezza della necessità di arrivare a regolamentare una professione

sicuramente non giova dal punto di vista dell'approfondimento del tema che si vorrebbe portare avanti, visto e considerato che il prodotto è questo. Quindi, si dimostra il contrario di quello che si vuole imporre col comma 2 di questo articolo. Pertanto, mi asterrò.

per le quali c'è un'esenzione da questo obbligo. Il suddetto comma 2 va letto congiuntamente all'articolo 19 di questo disegno di legge, che riguarda la sospensione dell'esercizio professionale. Per evidenti motivi, sui quali non mi dilungo, si è ritenuto di proporre che siano sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica i vertici istituzionali, e cioè il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e alcune altre categorie tra cui i membri della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura. Noi proponiamo che anziché esonerare totalmente, così come fa il comma 2 dell'articolo 10, categorie molto ampie di avvocati dall'obbligo di curare costantemente e continuamente il loro aggiornamento - una proposizione del genere da parte della maggioranza costituirebbe una sorta di privilegio a favore, ancora una volta, della casta dei politici, degli avvocati politici in particolare - si operi una limitazione di questa esenzione, nel senso che riteniamo che sia più opportuno che vengano esentati dall'obbligo solo coloro

e gli studiosi che hanno direttamente, giornalmente, a che fare con le materie giuridiche, quindi docenti e ricercatori confermati dell'università. Al di fuori di queste categorie è assolutamente incomprensibile - salvo che per volontà di creare un altro privilegio alla "casta" - un'esenzione dall'obbligo di aggiornamento. Non a caso, questo tema è stato riproposto anche in altri emendamenti, ad esempio nel successivo emendamento 10.217

tutti i presidenti di Provincia e tutti gli assessori provinciali, tutti i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. C'è un rispetto dovuto ai vertici istituzionali, ma non allarghiamo il numero di coloro che dovrebbero beneficiare di questo esonero. Un'ultima considerazione: siccome crediamo fortemente come Partito Democratico nella necessità di questa formazione e di questo aggiornamento continuo e costante, ricordo che - lo vedremo tra poco - con un emendamento successivo noi prevediamo delle garanzie di accesso, eventualmente anche con sostegno economico, a tutela di tutti coloro - penso in particolare ai giovani avvocati - che hanno interesse e volontà di partecipare a questa formazione continua. In conclusione, voteremo per la sostituzione

dei destinatari della sospensione dall'esercizio della professione; il problema è o di aumentare a dismisura l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio della professione, oppure di trovare un punto di equilibrio. L'articolo 19 estende notevolmente i casi di sospensione rispetto alla normativa attuale (la legge n. 215 del 2004, che prevede le incompatibilità e, quindi, la sospensione); però riconoscere che lo svolgimento di funzioni amministrative delicate in strutture amministrative di una certa importanza completamente se quelle funzioni amministrative rese nell'interesse della collettività devono essere assolte. Ritenere che l'assolvimento di queste funzioni delicate enti territoriali importanti sia compatibile con l'esistenza di un obbligo alla formazione continua significa imbattersi in una forma d'ipocrisia:

lo svolgimento di funzioni di amministratore deve comportare la sospensione di tali obblighi, ma non potevamo aumentare a dismisura la platea della sospensione; abbiamo cercato di trovare un punto di equilibrio su interessi tutti tutti meritevoli di tutela. È un punto di equilibrio ottimale? Speriamo. Qualora si realizzerà in futuro che il punto di equilibrio va corretto, il Parlamento sarà in grado di farlo.

venticinque anni di iscrizione all'albo, ovvero dopo il compimento del sessantesimo anno di età».

del Partito Democratico, vorrei sviluppare alcune riflessioni di carattere generale sulla natura della formazione permanente e sulla sua funzione, che va analizzata al di fuori di schemi lineari e convenzionali, come invece fa il disegno di legge e come fa, ancorché in qualche misura migliorandolo, la norma indicata nell'emendamento. Tutti gli studiosi dell'apprendimento e della formazione insegnano (è sufficiente consultare un semplice manuale di pedagogia) come il depauperamento delle capacità tecniche, delle informazioni (quello che viene chiamato analfabetismo di ritorno) si accentui, piuttosto che attenuarsi, nella fase della vita più avanzata.

che implica qualche maggiore difficoltà di gestione quanto più l'età avanza. È dunque sbagliato e contraddittorio, a nostro parere, prevedere un'esenzione dalla formazione permanente proprio dei soggetti che di questa formazione permanente, dal punto di vista delle conoscenze tecniche e degli strumenti per gestirle, avrebbero più bisogno. che è un'idea antica - come purtroppo lo sono molti elementi di questo disegno di legge - secondo cui il fatto di diventare più anziani, e quindi probabilmente più saggi, implichi anche un miglior controllo delle conoscenze tecniche. È esattamente il contrario. Si dovrebbe, semmai, prevedere un incremento dei meccanismi di formazione per gli avvocati più anziani, sia dal punto di vista meramente anagrafico che dal punto di vista degli anni di esercizio della professione. Molte cose si danno per scontate quando si fa un lavoro da tanto tempo e non si è sottoposti al vincolo del controllo periodico di professionalità; molte cose vengono considerate ovvie, quando ovvie non sono più, perché la tecnologia cambia, perché cambiano le norme e perché cambia il modo di interpretare, gestire le norme ed esercitare la professione come derivante dal connubio e dall'intersezione fra tecnologia, appunto, e norme stesse. Per tutte queste ragioni, pur consapevoli del fatto che l'emendamento in qualche misura riduce il negativo impatto della norma così come originariamente era stata concepita, dichiariamo il nostro voto di astensione.

Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto statale comprensivo «Mandes» di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, ai quali diamo il benvenuto.

Signora Presidente, capisco il parere contrario del relatore. È evidente, collega Valentino, che bisogna porsi la domanda di che effetto fa ai cittadini e ai colleghi avvocati - ormai 230.000 - leggere che gli avvocati che sono seduti in questo Parlamento sono esclusi dall'aggiornamento professionale che per tutti è richiesto

come anche i colleghi dell'opposizione si stanno comportando su questo provvedimento, non ne faccio un vanto - questa è proprio la cosa che fa vedere noi parlamentari come la «casta» invisa e odiata. odiata. È una di quelle cose semplici, collega Valentino, e mi rivolgo anche a voi, colleghi della maggioranza, al collega Longo che prima è intervenuto, provando a spiegare la sua opinione in materia. La giurisprudenza va avanti. Volete per caso dirmi che tutti gli avvocati che sono seduti nella Camera e nel Senato, oggettivamente, leggano tutti gli atti che questo Parlamento produce? Che lo dobbiamo presumere, è vero, collega Longo; tuttavia, collega Valentino, lei m'insegna, essendo più saggio e più esperto di me, che ciò non

e, cioè, esclude tutti i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, tutti i consiglieri regionali, tutti i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali, tutti i sindaci e gli assessori di Comuni sopra i 100.000 abitanti, e cioè quelli più in vista nel Paese. Vi rendete conto che, lasciando questa norma, diamo mano libera alla critica nei confronti della «casta»? «casta»? So benissimo quanto costi ai colleghi che sono seduti in quest'Aula, nella Camera e negli altri consessi indicati in questa parte del comma 2 dell'articolo 10 fare aggiornamento professionale; lo so, perché lo faccio anch'io, collega Valentino, e devo dirle, proprio perché ormai ci diciamo da sempre le cose come stanno - non è piacevole quello che sto per dire, collega Longo molti colleghi lo fanno ma, in realtà, non ci vanno, perché c'è qualcuno negli ordini che timbra loro qualcosa (vedo qualcuno che è assente dentro i banchi della maggioranza). È onesto ammetterlo, perché è così! così! Non è una pressione o una forzatura di colui che vi sta parlando. Allora, se è così, la giurisprudenza va avanti per i parlamentari, per i consiglieri regionali e per tutti gli altri soggetti indicati. Noi dobbiamo provare o concorrere ad eliminare dalla testa di molte persone nel nostro Paese l'idea che facciamo norme a tutela di questa casta e si può cominciare proprio

se non verrà approvata, darete al Paese la sensazione che per i parlamentari e la politica vi è una legge diversa da quella che si applica a tutti gli altri 229.000 avvocati italiani. Non v'è chi non veda che è così. compiere uno sforzo per mandare un messaggio diverso al Paese, molto più comprensibile e trasparente. Presidente, comprendo lo spirito che anima il collega Lusi e condivido le sue preoccupazioni rispetto al tema ricorrente dei vantaggi dei quali la «casta» sarebbe beneficiaria; la ragione sostanziale che ci ha indotto a confezionare questo articolo, d'intesa - lo ripeto sempre perché è bene che venga sottolineato - con i rappresentanti istituzionali dell'avvocatura e con tutte le associazioni di categoria,

significa che noi per primi abbiamo un po' perso la consapevolezza del ruolo che stiamo ricoprendo. Noi non svolgiamo un ruolo che può essere identificato con la «casta» e con il privilegio; noi siamo al servizio del Paese, cosa che comporta certamente dei sacrifici, e molti degli avvocati che siedono in questi banchi hanno fatto tantissimi Se, però, il meccanismo legislativo passa attraverso queste Aule, lei non vuole presumere che un minimo di aggiornamento anche sedendo tra questi banchi si possa fare? Noi siamo detentori per primi dell'innovazione legislativa:

di svolgere il loro ministero nelle aule di giustizia allorquando ciò sia possibile e compatibile con i numerosi e gravosi impegni che il compito parlamentare impone; nello stesso tempo dobbiamo anche immaginare

Probabilmente nel suo mandato avrà a che fare molto di più con questioni legate all'amministrazione, magari molto più complicate che andare a rappresentare alte cariche dello Stato nelle aule dei nostri tribunali. In ogni caso, non credo abbia assolutamente il tempo di poter mantenere al livello necessario la propria preparazione professionale. Pertanto, mi astengo su questo emendamento.

chiedo anche a lei, che appartiene al ceto forense, se ci stiamo prendendo in giro. Qualsiasi avvocato sa benissimo che l'aggiornamento professionale, per cento in un aggiornamento riferito alle novità giurisprudenziali e dottrinali e solo per il 5 per cento o anche meno sulle novità legislative. Quello che si chiede all'avvocato, e che è particolarmente oneroso per l'avvocato che vuole servire bene il proprio cliente, è conoscere tutte tutte le novità giurisprudenziali, come l'ultima sentenza di Cassazione, magari non ancora pubblicata su una rivista e che, però, può servire per vincere la causa. La novità legislativa incide su questo onere di aggiornamento in misura minima, anche perché è molto più facile conoscere la nuova legge che non conoscere l'ultimo grido della giurisprudenza o della dottrina. Ora, se questa è la vera materia di cui stiamo parlando, veramente non riesco a capire come si possa sostenere decentemente che un assessore regionale o un consigliere regionale, come anche un parlamentare, si aggiornino sulla giurisprudenza e sulla dottrina per il solo fatto di sedere in un consiglio comunale o in un'Aula del Parlamento. È veramente una presa in giro di cui dobbiamo fare giustizia. è dunque evidente che le norme delle quali stiamo discutendo costituiscono soltanto una esenzione per la casta dei politici, rispetto a un onere di cui vogliamo caricare soprattutto i più giovani. Di fatto, quest'onere graverà soltanto su quelli che escono dall'università e sui loro primi quattro anni di professione.

anche alla riformulazione richiesta dal relatore al senatore Caruso. Lei ha detto, invece, che il parere era contrario e quindi si sono invertite le parti. Ora, indipendentemente dall'incidente di percorso, che può sempre sembra di capire che, comunque, tutta la tensione necessaria per concludere l'*iter* di questo provvedimento non esista. Io mi domando allora se sia il caso di continuare in questo modo ad affrontare una questione fondamentale come la riforma di un ordine professionale.

Signor Presidente, con l'emendamento 10.221 mi ero proposto di semplificare la vita, per dirla in maniera a coloro i quali nelle Regioni hanno responsabilità di governo, quindi gli assessori regionali, e mi era sembrato fosse superflua la disposizione con riferimento ai consiglieri regionali.

che viceversa, se avessi ben compreso, avrei votato a favore. Ora, tuttavia, disposto come sono a ritirarlo, le chiedo per quale ragione sia precluso l'emendamento 10.224, che si riferisce agli assessori provinciali. Credo che nella pletora di coloro che sono esentati non debbano essere compresi gli assessori provinciali.

Si dicono tante cose - se lei sapesse quante! - che suscitano ilarità, e da tempo lontano!

E sappiamo tutti che un buon avvocato fa ottimamente gli interessi della giustizia in generale. Quindi, il fatto che si lasci unicamente al Consiglio nazionale forense la possibilità di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, lasciando completamente fuori il Ministro della giustizia,

Direi di votare per parti separate.

nei confronti del quale nutrivo alcuni dubbi in relazione ad alcune parti che non riguardavano, tuttavia, quello su cui si è incentrato il parere contrario della 5a Commissione e che ha condotto alla sua reiezione.

L'emendamento 10.232, pur trattando lo stesso tema, dice una cosa assolutamente contraria: i consigli degli ordini non possono tenere dei corsi di formazione a titolo oneroso. Quindi, l'emendamento apre due vie: o i consigli degli ordini non tengono non tengono corsi di formazione, perché non possono farlo senza risorse, oppure trovano risorse nell'ambito dei propri bilanci, o meglio, all'esterno dei propri bilanci, ad esempio attraverso sponsorizzazioni. L'emendamento aggiunge che i consigli degli ordini non possono patrocinare enti esterni che a titolo oneroso prestino servizi di formazione,

La invito, signor Presidente, ad accantonare questo emendamento e a chiedere alla 5ª Commissione di riesaminare la questione e di voler modificare il proprio parere, o, in alternativa, di indicare quali sono le risorse pubbliche sensibili al parere della 5ª Commissione che vengono toccate da questo emendamento che impartisce semplicemente una disposizione: i consigli degli ordini, se non hanno i soldi all'interno del proprio bilancio, non possono tenere corsi di formazione a titolo oneroso. Credo che sia un problema molto delicato, signor Presidente, perché a fronte dell'affermazione politica che non si impongono nuove tasse, in realtà, se imponiamo ad una serie di cittadini l'obbligo, affinché possano esercitare il loro diritto primario a svolgere un lavoro, di praticare dei praticare dei corsi a titolo oneroso, nella sostanza facciamo proprio quello che in altri luoghi diciamo di non voler fare.

Vorrei far presente soltanto un aspetto. Sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Caruso. Si tratta della prima questione che ho sollevato sul primo emendamento che abbiamo trattato. Vi è stato, però, un rifiuto di accantonamento.

solo per chiarire un punto, signor Presidente, per l'esistenza di un principio di carattere generale. Esiste un elenco delle pubbliche amministrazioni, quale non comprende soltanto le amministrazioni pubbliche in senso stretto, ma anche gli organismi - gli ordini professionali fanno parte di detto elenco - che svolgono attività di interesse pubblico. Per questa ragione, quindi, esiste un interesse pubblico a tutelare l'equilibrio dei loro bilanci. Mi riferisco - per esempio - alle casse previdenziali completamente private, il il cui *default* determinerebbe sul bilancio pubblico effetti molto negativi qualora lo Stato si dovesse trovare - e si è già trovato - nelle condizioni di dover intervenire quando la cassa previdenziale completamente privata non è in grado di soddisfare agli impegni assunti con coloro che hanno contribuito. Risultato: gli ordini professionali - non perché la 5a Commissione lo voglia o no - fanno parte di questo elenco. Ne consegue che qualsiasi ipotesi di intervento di spesa a carico di questi enti deve essere sottoposta ad una valutazione particolarmente severa poiché fanno parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni. Organizzano i corsi, ma li pagano quelli che vi partecipano: se li paga qualcun altro, cioè l'ordine, è del tutto evidente che questo va a carico di una finanza pubblica allargata così come risultante dall'elenco delle pubbliche amministrazioni. Non è un parere, è un fatto. È un fatto estremamente delicato quello che lei pone, sempre con la dovuta competenza ed arguzia. Mi auguro che la 5a Commissione possa affrontare il tema. Lei, senatore Morando, ci ha già posto un'ampia

ci sono numerosissime soluzioni a questo problema. Per esempio, si può stabilire che coloro che sono in grado di pagare per frequentare i corsi paghino una quota aggiuntiva rispetto al costo individuale del corso per fare fronte al costo della partecipazione al corso di persone che non possono pagare. Una cosa è sicura, però: non si può dire per legge

Nell'ambito delle soluzioni che prevedano che i soggetti che partecipano al corso paghino, naturalmente si possono fare delle esenzioni, condizione che coloro che sono in grado di farlo partecipino più di quanto sarebbe necessario per coprire i rispettivi costi, in maniera da coprire i costi relativi ai soggetti che non possono pagare.

Signor Presidente, io sono di prima nomina, quindi magari non m'intendo di lavori della nostra Assemblea, ma mi pare di essere in fase consultiva. È arrivato un disegno di legge. Tutti esprimono il proprio parere relativamente alle norme che non hanno a questo punto mi viene di dire - trovato consenso in Commissione. Si apre un dibattito in cui ci si toglie la propria veste istituzionale e si partecipa con dei contributi a migliorare un testo che, sinceramente, ha ancora bisogno di un grande lavoro:

al merito vorrebbero in effetti un'ulteriore sospensione di approfondimento - mi

nella tematica, perché non vi è dubbio che gli ordini facciano parte di quell'elenco. Vorrei fare però presente che una delle soluzioni prospettate,

che, a prescindere da ogni altro rilievo, oggettivamente almeno le somme necessarie per partecipare ad un corso di formazione debbono averle. Diverso potrebbe essere per il praticante avvocato, e potrebbe essere un'altra forma di ragionamento, ma in questo caso credo che quel tipo di soluzione prospettata, che potrebbe avere una sua logica sarebbe francamente forse non applicabile.

è un termine che va precisato, perché le cose sono gratuite per chi ne usufruisce, ma chi le produce ne ha un onere. Nel caso specifico, per tornare all'apprezzabile intervento del senatore Morando, l'onere è affrontato dal soggetto pubblico che, in questo caso, è l'ordine professionale. Allora, la gratuità che determina sicuramente un intervento di natura sociale apprezzabile, condiviso, assolutamente giusto e corretto - deve essere bilanciata a favore di chi quella gratuità ha prodotto affrontando un costo. Chiunque consuma un piatto di pasta gratuitamente deve sapere che quel piatto qualcuno l'ha prodotto e per produrlo ha affrontato un costo;

che lo si faccia per tutta la legge. Lo dico per evitare che la 5a Commissione faccia la parte del «signor no», quando non ne ha nessuna intenzione e soprattutto non ha nessuna competenza in relazione al merito.

alle garanzie di accesso, alla formazione e alla specializzazione di avvocati. Io credo che in tutto il corso della discussione di questo importante disegno di legge abbiamo sempre avuto in grande considerazione le condizioni economiche di chi accede a questa professione, proprio per non dare luogo a discriminazioni o a impari opportunità,

ha appena iniziato, e questo forse sarà compito di un regolamento del CNF, ma io credo che così, *tout court*, pensare di

sulla natura giuridica dei consigli dell'ordine, a me consta che sono enti pubblici non economici: questa è la definizione che mi pare di dover sostenere. Presidente, vorrei sottoporre ai colleghi della Commissione bilancio un precedente. In occasione dell'aumento dell'ambito di competenza del giudice di pace, la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo ritenendo che tale aumento potesse determinare un lavoro in più e quindi una retribuzione in più. In realtà, così non fu perché il *plafond* che era stato fissato non poteva comunque essere superato. Analogamente, in questo caso si è fissato un *plafond* di contribuzione per un consiglio dell'ordine che viene equiparato all'ente pubblico. La circostanza che il Consiglio dell'ordine debba sopportare un onere aggiuntivo non significa necessariamente sforamento del *plafond*: significa riorganizzare le risorse anche alla luce del compito aggiuntivo. Quindi, non riesco a comprendere, anche naturalmente per mia deficienza di conoscenza dei bilanci, tali obiezioni. Presidente, considerata la sua attenzione e anche la disponibilità ad accogliere come ricevibile le finalità di questo emendamento e avendo trovato come unico ostacolo quello relativo alla Commissione bilancio, che ancora sul merito non si è pronunziata, vorrei ricordare che probabilmente - lo dico a beneficio anche dei lavori di approfondimento che la Commissione bilancio svolgerà nelle prossime ore prossime ore - l'emendamento potrebbe trovare un più facile accoglimento se si eliminasse la parte relativa alla cassa nazionale di previdenza. Come Come osservava anche il senatore Morando poc'anzi, le casse di previdenza sono sottoposte agli obblighi della finanza pubblica, perché sono fondazioni di diritto privato. sono esclusi dall'elenco che annualmente l'ISTAT redige, nel quale vengono inserite tutte le amministrazioni pubbliche sottoposte all'obbligo del rispetto del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente gli ordini professionali, come ricorda anche il Sottosegretario, pur essendo enti di diritto pubblico non economico, non devono sottostare agli obblighi previsti per gli enti inseriti in questo elenco indicato dal riferimento normativo che ho poc'anzi detto, nel quale invece rientrano le fondazioni relative alle casse di previdenza. Conseguentemente, credo che il principio di garantire l'accesso all'attività formativa a titolo non oneroso ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio possa essere tranquillamente attribuito al bilancio di ciascun ordine; ciò infatti non determina dei problemi di tenuta economica, sia per i motivi ricordati poc'anzi dal senatore sia perché gli ordini professionali, torno a dire, ancorché enti di diritto pubblico, non sono sottoposti agli obblighi del rispetto del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

il parere stesso. Cioè, si disquisisce sulla natura giuridica delle associazioni professionali: enti pubblici, enti pubblici non economici, eccetera. Il quesito che si pone alla Commissione bilancio, come è stato già detto, è

perché sono comprese in quell'elenco? Perché lo Stato si è preoccupato, poiché svolgono funzioni di carattere pubblico, che una loro cattiva gestione finanziaria determini un onere aggiuntivo nel futuro. L'esempio della cassa previdenziale è, naturalmente, quello più facile da fare, anche perché in quel caso il

però l'abbiamo già svolta approfonditamente ed abbiamo concluso che se i partecipanti al corso pagano il costo dei corsi non c'è problema; se invece si vuole affermare che per loro è gratuito, allora bisogna trovare un'altra copertura. Non è possibile affermare che si svolge un'attività di questo tipo per obbligo di legge

all'origine che questo ordine debba diventare pubblico e stabiliamo che, visto che dobbiamo tagliare la spesa di decine di miliardi, ce ne accolliamo ancora un'altra fetta, ciò diventa un problema, e non siamo d'accordo. Viceversa, se la questione rimane nell'alveo del privato, non c'è alcun problema: questi corsi verranno pagati dagli avvocati e dagli associati.

i corsi di aggiornamento si svolgano periodicamente e qualitativamente in maniera apprezzabile, si auspica poi che si possa realizzare anche un sostegno economico per quelle per quelle categorie e per quelle aree della professione che non siano in condizioni di affrontarne gli oneri.

coloro i quali non sono in grado di sostenere questo costo, lo vedranno sostenuto da una maggiorazione dell'impegno finanziario al quale saranno soggetti gli altri avvocati: quasi un fondo di accantonamento a costo zero. Possono essere tante le soluzioni.

l'emendamento 11.200, facendo seguito a quanto lei ha appena detto, con la speranza di trovare una condivisione di principio su quello che poco fa il rappresentante del Governo ha voluto chiamare impari opportunità. L'articolo 11 parla di assicurazione e responsabilità civile; lo leggo perché credo che il clima odierno necessiti di pause di ulteriore approfondimento della materia che stiamo affrontando. «L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa».

a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Quindi, si chiedono avendo a che fare con documenti sensibili e di grande importanza per lo svolgimento della professione stessa e sapendo che all'interno degli studi legali agiscono anche

e nelle mani del fato, che potrebbero creare problemi successivi di responsabilità civile per quanto riguarda l'avvocato. Conseguentemente, vorremmo sostituire la rubrica con la seguente: «Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni».

anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Quindi, si chiedono ulteriori modifiche dal punto di vista testuale, in particolare adottando, al comma Nella fase del dibattito generale, il relatore ha affermato che non si possono estendere ai cosiddetti praticanti alcune norme che invece vengono previste per chi fa già parte della professione, perché il praticante in qualche modo si

tale motivazione possa essere condivisibile, non credo che possa essere estesa, dal punto di vista delle assicurazioni degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, con un approccio di questo tipo. Quindi, chiediamo che debba debba essere stipulata anche un'assicurazione per gli infortuni nei confronti dei collaboratori.

come ipotizzano gli emendamenti, o alla mera facoltà su richiesta, come ipotizza il testo del disegno di legge, di rendere manifeste la sussistenza della polizza assicurativa ed i suoi estremi. In realtà, la questione, nella sua apparente minuzia tecnica, investe un profilo fondamentale del rapporto fiduciario tra il cliente e l'avvocato. Cerco di spiegarmi in modo lineare. Nel momento in cui si crea il rapporto e l'incarico viene affidato, si verifica dal punto di vista psicologico, oltre che dal punto di vista giuridico, un affidamento importante di un soggetto nei confronti dell'altro. la scelta dell'avvocato è un'operazione che ha molto a che fare con una dimensione psicologica di fiducia personale, oltre che con profili più tecnici inerenti alla specializzazione e dunque alla competenza del professionista. polizza vengano resi noti solo a seguito di una richiesta del cliente implica sostanzialmente uno svuotamento della norma, perché in quella fase delicata dell'affidamento dell'incarico e dell'affidamento, per molti aspetti, della propria persona e del proprio destino, è fortemente improbabile che il cliente rivolga la richiesta formale all'avvocato di comunicargli la polizza e i suoi estremi. Vi è una sorta di antitesi psicologica tra l'affidamento e la richiesta, il cui contenuto e la cui premessa hanno carattere di sfiducia metodica, degli estremi relativi alla polizza. È uno di quei tipici casi, come accade in tantissime altre

in cui è indispensabile un automatismo, proprio per evitare i negativi effetti psicologici e quindi il sostanziale svuotamento della facoltà che deriverebbe dall'esercizio pratico

si prevede che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare una polizza assicurativa.

ho registrato l'intento unanime, una volta che si sarebbe tornati su questo tema, di incardinarlo in Aula per andare avanti fino alla sua definizione. In tal senso vi è stata una convergenza. i tempi non erano stato disciplinati, ma io sono dell'idea che, per mantenere fede a questo impegno condiviso da tutti,

dell'Assemblea e riguarda una riforma importante quale quella della professione forense, si era convenuto - e credo che il senatore Zanda lo ricordi bene, e del resto il suo dire di adesso non contraddice

vuol sapere quali sono le decisioni, e questo mi sembra legittimo. Si convenne di non procedere ad un contingentamento rigido dei tempi perché c'era la volontà di arrivare alla conclusione.

tra alcuni provvedimenti ed altri. Spesso ci si lamenta dei decreti, dei tempi contingentati e dei voti di fiducia: questa volta stiamo discutendo un provvedimento che è frutto delle iniziative parlamentari senza voler soffocare la discussione; deve anche avere un punto di approdo e mi auguro che domani, al termine della seduta antimeridiana, si possa definire un percorso.

un atto politico del Ministro della giustizia, compiuto al Congresso nazionale forense di Bologna di due anni fa. A nostro avviso, le difficoltà che sta incontrando questa riforma in sede di discussione in Parlamento non sono casuali, ma nascono da un difetto di impostazione: l'avere cioè assunto come unici come unici interlocutori del potere legislativo nell'impostazione della riforma gli avvocati, quando invece la disciplina della professione ha come principale referente, principale soggetto interessato l'amministrazione della giustizia, e poi gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori, i quali sono stati invece tenuti totalmente fuori dall'itinerario di formazione di questo testo legislativo; tanto che, per esempio, elementari principi di tutela della concorrenza sono totalmente obliterati, pretermessi. Chiedevo stamattina e torno a chiedere che, prima ancora che si riunisca la Conferenza dei Capigruppo, il Governo ci dica se rispetto a quella impostazione iniziale c'è una modifica nel suo intendimento riguardo a questa riforma oppure no;

un quadro definito, nella certezza di venire incontro alla volontà di tutti i Capigruppo quando hanno deciso di riportare il testo in Aula per arrivare al voto finale.

sono aggiornati ogni cinque anni».

«Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati

richiama lo spirito di concordia e collaborazione nell'affrontare un tema così delicato. È vero: questa riforma è cominciata addirittura nella scorsa legislatura, forse molto prima, ma vi abbiamo lavorato seriamente e vogliamo che abbia uno sbocco.

agli avvocati, questa polizza deve seguire un *iter* e deve avere delle caratteristiche in funzione di garanzia. Gradirei che il relatore Valentino mi ascoltasse, perché ho fiducia nella sua sensibilità.

perché, visto che l'assicurazione è una previsione condivisa e obbligatoria nell'interesse dell'utente? Non voglio ripetere quello che ha detto poco fa il collega Ichino tentando di riportare l'Assemblea a questo punto, veramente

entrino in vigore contestualmente, secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione; tuttavia non è possibile subordinare l'entrata in vigore di un atto normativo ad un altro atto ancora da emanare, peraltro in un'altra autorità come quella europea. Inoltre, la normativa europea si applica nell'ordinamento interno in virtù di meccanismi di recepimento che non possono essere disciplinati o alterati

l'assicurazione, la quale ha a che fare in ultima istanza con la responsabilità civile dell'avvocato. infatti, che nell'esercizio delle funzioni l'avvocato si avvalga di collaboratori in pianta stabile o occasionale, i quali possono avere una serie di problemi di vario tipo, genere e natura, durante lo svolgimento delle loro funzioni. funzioni. Il fatto di tutelare queste persone in qualche modo credo vada a rafforzare anche la tutela dello stesso avvocato relativamente alla sua responsabilità civile, in particolare ove si ritenga di doverla ampliare anche ai documenti che sono al centro della sua attività lavorativa. Come già detto, si sa che non è l'avvocato in persona che maneggia tutto ciò, ma sono i suoi collaboratori. Qualora dovesse accadere qualcosa a questi ultimi, la responsabilità finale sarebbe sua, ma tutelare anche chi lavora per lo scopo finale della professione potrebbe essere utile. Vorrei poi chiosare una dichiarazione poc'anzi resa dal senatore Maritati. Non stiamo ora facendo una riforma per il miglior funzionamento della giustizia. La riforma della giustizia, più volte auspicata, proclamata e annunciata dalla maggioranza la dobbiamo ancora vedere. Qui si tratta di regolamentare una professione, ampliando moltissimo i poteri dell'ente che poi ne dovrà tenere conto. Sicuramente i problemi della giustizia in Italia, che sono

emendamento che trattasi certamente di una legge diretta a regolare il settore dell'attività forense, che riteniamo essenziale ad un corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Mi sorprende che anche il collega Perduca sia caduto in questo equivoco, che ritengo pericoloso. Anche nel momento in cui abbiamo affrontato l'ordinamento giudiziario non era qualcosa che riguardasse solo i magistrati: riguarda immediatamente i magistrati, ma perché vi sia un funzionamento più all'altezza dei compiti, e quindi al fine di garantire un corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Questa legge è importantissima perché l'avvocatura è uno dei pilastri del sistema dell'amministrazione della giustizia. Non è possibile sperare che funzioni bene, finalmente, questo settore vitale della vita sociale e pubblica, nostro Paese, se anche gli avvocati non si attrezzeranno, se anche l'avvocatura non avrà le riforme per le quali stiamo lavorando. Quindi, su questa premessa, insisto anche per l'accoglimento dell'emendamento dell'emendamento 11.210, perché non comprendo, trattandosi di un settore molto delicato quale quello della polizza assicurativa, perché non debbano essere sentiti altri organi di vitale importanza per il corretto funzionamento di questo aspetto particolare e di tutto il complesso dell'attività giudiziaria. [LI Stiamo parlando di rendere obbligatoria una assicurazione per la responsabilità civile risultante dall'attività professionale. Non capisco, ai fini ai fini dell'assicurazione per la responsabilità civile, cosa ci possa entrare il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione. Stiamo

che ritenevamo necessario introdurre per modificare in senso migliorativo la norma è - mi si passi l'espressione - metafora dello spirito stesso della norma, nel momento in cui si introduce un elemento che mira, in termini di sistema, oltre che sotto un profilo specifico e tecnico, a ridefinire in meglio, nel senso di una maggiore trasparenza e di migliori garanzie, il rapporto tra il cliente tra il cliente e l'avvocato. È necessario essere consapevoli, come ho detto in precedenza, dei delicati profili psicologici che caratterizzano questo rapporto, anche e soprattutto nella fase introduttiva, in cui si genera quella peculiare relazione che poi genererà - mi si passi l'espressione tecnica, un po' quel litisconsorzio necessario prolungato nel tempo tra cliente e avvocato. Pensiamo alla pratica quotidiana, non ragionando su categorie astratte: pensiamo al cliente che per delicate vicende che coinvolgono la sua sfera, a volte intima, si rivolge all'avvocato, in sede penale o anche civile, in quegli ambiti in cui più pro,fonda è la penetrazione del diritto nella vita privata: pensiamo alle vicende matrimoniali, alle vicende che riguardano i minori, a tutte le vicende in cui il soggetto - sia egli persona offesa o indagato - si rivolge all'avvocato per chiederne l'assistenza nella sede penale. In tutte queste vicende è improponibile e inimmaginabile che il cliente chieda all'avvocato di fornirgli informazioni che sono psicologicamente e concettualmente incompatibili

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'auspicio, la richiesta che il Popolo della Libertà fa di accelerare al massimo e di condurre a compimento quest'atto non ci esonera dall'opportunità di sottolineare con forza la grande portata di questa norma, che a taluni può apparire quasi scontata, ma non lo è affatto. Si tratta di introdurre un obbligo che fino ad oggi non sussisteva nel nostro ordinamento, ordinamento, e per un verso sono contento che una volta tanto anche con il collega Maritati e con l'opposizione ci si trovi d'accordo sul fatto che questa non è esclusivamente una norma posta a difesa o ad interesse esclusivo della categoria e della professione forense ma si inserisce appieno nella multiforme necessità che funzioni bene il mondo della giustizia, delle cause, dei processi, del rapporto tra professionista e cliente, che poi in definitiva il soggetto a cui sempre dobbiamo guardare, nel suo interesse, nell'interesse del buon funzionamento della giustizia. Quindi, stiamo lavorando ad una riforma che è ingranaggio essenziale della riforma complessiva della giustizia. Aggiungo che questa norma assolutamente virtuosa che stiamo inserendo e prevedendo per la prima volta nel nostro ordinamento testimonia anche, se vi fosse stata qualche preoccupazione, che non stiamo affatto con la nostra iniziativa adagiandoci esclusivamente su un interesse categoriale o egoistico degli esercenti la professione forense: stiamo tutelando il cliente ed il cittadino, il detentore e il portatore di diritti, e stiamo cercando di far sì che ogni sfasatura, ogni inconveniente, ogni errore, ogni colpevolezza

oneri per la formazione professionale, resa obbligatoria e continua, e oneri per la polizza assicurativa al fine di rispondere al cliente. Mentre noi stessi, convinti fautori di questa legge, reclamiamo per il ceto forense responsabilità, dignità, ed anche tutele e rafforzamento del proprio ruolo, opponendoci a norme che lo vadano a penalizzare, nello stesso tempo, correttamente, vogliamo un rafforzamento degli obblighi deontologici, e anche economici ove occorra, perché la professione, sia a livello di diritti, di poteri, di responsabilità e di ruolo, ma anche di doveri, si innalzi nel suo livello. Direi quindi che con soddisfazione, registrando che perlomeno non vi sono voti contrari, sottolineiamo l'innovatività, l'importanza e la virtuosità di questa norma che approviamo.

l'articolo 12 del disegno di legge si occupa delle tariffe professionali, cioè di una di quelle questioni che, come non mai, sono state solo oggetto di mistificazione. La massima parte degli avvocati, a quattro anni di distanza dai provvedimenti del Governo di centrosinistra sul tema, mostrano ancora di non aver digerito la novità della rimozione dei minimi tariffari dalle loro tariffe e dell'abrogazione del divieto dei patti di quota lite. Dall'altra parte, continuano ad affaticarsi sulla questione almeno due importanti centri di opinione, vale a dire, in primo luogo, gli imprenditori, e per essi la loro massima associazione, cioè Confindustria, e, in secondo luogo, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Gli imprenditori Gli imprenditori hanno sempre avuto, nei confronti dei professionisti, sentimenti assolutamente opposti e contrastanti, al limite del surreale: li hanno in odio quando sono loro fornitori, detentori di saperi di cui non è possibile fare a meno, e quindi quando chiedono, come tutti i fornitori, il controvalore delle prestazioni che rendono (insomma, li hanno in odio quando presentano parcelle alle loro imprese); li amano molto tutte le volte che tentano - ormai il fatto è risalente e ricorrente - di appropriarsi dei loro saperi per farne prodotto d'impresa, oltre che per impossessarsi della loro indipendenza. Sto parlando delle risalenti e ciclicamente ricorrenti proposte di aprire l'esercizio dell'attività professionale (dell'avvocato, in questo caso) alle società di capitali e quindi di fornire prodotto nuovo a chi vuol fare impresa, ovvero nuovo *business* a chi già fa impresa: alle grandi società, ai grandi gruppi, con il non celato fine - tante volte - di rivitalizzarne conti tendenti a divenire traballanti quando generati dalle produzioni tradizionali. I Governi di centrosinistra sono stati sensibili alle suggestioni di vario genere a sostegno di tale idea. Lo sbarramento posto in essere dai professionisti finora ha retto. In futuro vedremo che succederà.

L'Autorità si è infatti schierata senza esitazione, su uno dei punti di vista comunitari in argomento, nella direzione di considerare le tariffe obbligatorie come causa di diniego di opportunità e di limitazione della concorrenza. Su uno solo dei coesistenti punti di vista comunitari - lo ripeto - perché è ormai palese che, in sede di governo europeo, è con grande disinvoltura che si giustificano plurime e discordanti opinioni tutte le volte che le questioni toccano più interessi molteplici. Ebbene, ecco dunque il comune denominatore argomentativo impiegato sia dagli imprenditori, sia dall'Autorità garante, che condusse l'onorevole Bersani, allora Ministro dell'industria del Governo Prodi, a "lenzuolare" (giusto per usare il neologismo allo allo stesso caro) l'obbligatorietà dei minimi tariffari abrogandola ed affermando che in tale maniera si sarebbero aperte alla concorrenza le prestazioni professionali, a tutto vantaggio dei consumatori. Minimi tariffari abrogati, dunque, e rimozione del divieto del patto di quota lite: un vero toccasana - a loro opinione - per la collettività dei consumatori. Non è affatto così e si tratta - come dicevo - di una mistificazione non ulteriormente sopportabile. In sé, nel caso degli avvocati, è semplicemente surreale parlare di mancanza di concorrenza quando lavorano in Italia (o cercano di lavorare) oltre 230.000 soggetti che quotidianamente si misurano fra loro:

per le ragioni che ho più volte esposto anche in quest'Aula e che sono (almeno in parte) ricadenti proprio su responsabilità attribuibili al mondo delle imprese. Ma al di là di ciò e accantonato quindi il risibile quanto suggestivo argomento della mancanza di concorrenza e del relativo danno ai consumatori, il punto è visibilmente un altro. Premesso che il principale problema per moltissimi dei 230.000 avvocati italiani purtroppo non è oggigiorno quello di non avere tariffe minime ma, semmai, quello di vedersele pagate, le dette tariffe,

un vantaggio enorme che va in danno dei professionisti e in danno, ancorché indiretto, dei consumatori. Darò lettura di una lettera di poche righe presa a caso, fra le tante che mi sono state fornite da avvocati, in quanto tutte uguali nella sostanza. Si tratta di una lettera scritta da una grandissima banca nazionale, che ormai si potrebbe definire un "concentrato" di banche, e diretta ad un'avvocatessa - permettetemi di ometterne nome e città di residenza - che opera nel Nord-Est, non conosco ed a cui ho parlato per telefono; una donna giovane che svolge la professione come tanti. Si tratta di una causa avviata dal curatore di un fallimento in cui è chiesto alla banca stessa di restituire 365.000 euro, oltre agli interessi, in sede di revocatoria. Ecco cosa scrive la banca: «Gentile avvocato, faccio seguito alle conversazioni intercorse e con la presente trasmettiamo atto di citazione notificato alla nostra banca. Le confermiamo la nostra disponibilità a conferire l'incarico per la difesa giudiziale di (...). Detto incarico è tuttavia condizionato all'applicazione, per l'attività che sarà da lei prestata, della convenzione già in essere con la nostra capogruppo, tenuto conto del valore della controversia che quantifichiamo convenzionalmente in euro 42.000», e non - aggiungo io - nei 365.000 euro rivendicati in sede di citazione.

L'avvocatessa, giusto per la cronaca, ha accettato l'incarico e l'Associazione degli avvocati di cui fa parte dovrebbe, quindi, senz'altro espellerla, quantomeno a sentire le lezioni di legalità che ci vengono di recente impartite. Non avverrà senz'altro (per fortuna), ma è del tutto chiaro che si tratta di situazioni non oltre tollerabili a cui occorre porre rimedio, intanto legislativo. Confido nel parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento 12.202 che affronta il tema da molteplici punti di vista, compreso quello della incondizionabilità dell'incarico dato all'avvocato, nella costruzione che ci è giunta dal lavoro svolto dalla Commissione giustizia con l'approvazione (mi riferisco in particolare al comma 5) degli emendamenti lì proposti. Presidente, non illustrerò gli altri emendamenti che ho presentato;

che, qualora dovesse essere approvato l'emendamento 12.202, lo stesso dovrà essere integrato con il riferimento

finestra"). Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo statale di primo grado «Roberto Bracco» di Napoli. Rivolgiamo a loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio.

«Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione

della libera concorrenza e della possibilità di prevedere un accordo tra il libero professionista e il proprio cliente. infatti a fissare per legge il fatto che esistono degli onorari minimi, che sono inderogabili e vincolanti, mentre poi si prevede che, se qualcosa può essere derogato, sono proprio i limiti massimi tariffari;

sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali».

nel mercato dei liberi professionisti e quindi degli avvocati. L'*Antitrust*, che si è espressa

possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi. Secondo i consolidati principi *antitrust*, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso. Infine, occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi. L'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari (esattamente quello che si propone con la norma in esame): il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale. L'Autorità ricorda che l'articolo 2233 del codice civile, pure richiamato nel comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro.

il parametro di riferimento al fine di determinare un «compenso ulteriore» da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti Con la riforma Bersani sull'abolizione dei minimi tariffari e sull'inserimento della possibilità di contrattazione di prezzi e preventivi, si era quasi creduto che finalmente qualcosa cominciasse a cambiare. si aprissero spazi per l'utente verso una maggior trasparenza in merito ai costi e agli accordi con il proprio legale. Il preventivo scritto, in ragione della normativa introdotta, forniva al cliente un valido strumento di programmazione dei costi e di bilanciamento con i relativi benefici, prima di affrontare un'azione giudiziaria,

alea e discrezionalità su quanto alla fine fatturare all'assistito. Occorre invece creare meccanismi di trasparenza che consentano a chi intraprende un'azione di forfetizzare grosso modo i costi della stessa, anche non modificando l'attuale

sulla protesta degli agricoltori e dei contadini che hanno dato vita ad una manifestazione che è andata ben oltre le loro pacifiche intenzioni. Pacifiche intenzioni che si sono tramutate in rabbia e quindi anche in scontri violenti contro le forze dell'ordine,

coinvolte, tra cui anche semplici cittadini che non partecipavano direttamente a tale manifestazione. Credo che tutti abbiano ascoltato quanto è avvenuto dagli organi di stampa e in modo particolare dai telegiornali. verificare quanta disperazione e quanta sofferenza c'era nelle parole di alcuni manifestanti che mettevano in rilievo lo stato di esasperazione e di disperazione profonda di chi non trova risposte nelle istituzioni ad un problema gravissimo

La Sardegna soffre ormai da troppo tempo per una situazione di distanza e superficialità con cui le istituzioni stanno regolando alcune questioni di estrema importanza e vitalità per la Regione stessa sotto il profilo economico economico ed anche della coesione sociale. Stabilimenti che chiudono, aziende multinazionali che se ne vanno nell'indifferenza totale del Governo, che non trova di meglio che non dare risposte, neanche a livelli minimali. Credo che questa situazione debba essere vigilata, soprattutto dal Governo, con una lente di ingrandimento che, sfrondando la superficialità con cui tali questioni sono state regolate fino ad oggi, vada ad intervenire in maniera costruttiva e positiva in questa Regione, dove la povertà ed anche la situazione di insularità stanno determinando un problema sociale cui non possiamo non dare risposte. Chiedo pertanto, anche a nome dell'intero

dopo aver svolto un accurato accertamento su quanto avvenuto, venga a riferire in Aula sia sull'accaduto, che sui provvedimenti che il Governo intende adottare per arginare questa pesante e difficile situazione, che può anche sfociare in qualcosa di peggio. la Presidenza prende atto del suo richiamo ad una vicenda di ieri che ha turbato tutti e che è di grande importanza, che lei ha bene rappresentato nei

Signor Presidente, la lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali è un elemento che sta nel DNA del Partito Democratico. È certo che grazie al duro lavoro di magistrati e forze dell'ordine, che non hanno a disposizione mezzi adeguati, sono stati assestati durissimi colpi a tutte le mafie, ma nonostante questo, su *input* del Ministero dell'interno, i Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica delle prefetture si sono riuniti per ridurre le scorte. Nel dovuto rispetto per il Comitato per l'ordine e la sicurezza della prefettura di Palermo, ritengo un errore aver declassato i servizi di scorta al senatore Lumia,

ad essere oggetto di intimidazioni, peraltro riscontrate dagli organi preposti. Ecco perché chiedo a lei di riferire al Presidente del Senato di invitare il ministro Maroni alla rivisitazione del provvedimento, invitandolo ad evitare l'uso del manuale Cencelli per l'attribuzione delle scorte con una sorta di «una a te, una a me» su un tema delicatissimo. Bisogna valutare oggettivamente caso per caso. Affido al buon senso del presidente Schifani l'intervento nei confronti del ministro Maroni.

il palazzo di Santa Maria in Aquiro, che ha una superficie totale di 3.000 metri quadri e dal quale un progetto prevede di ricavare 51 uffici. La ristrutturazione è costata 25 milioni di euro, di cui 20,5 finanziati dal Provveditorato alle opere pubbliche e 4,5 dal Senato. Ogni anno il Senato, da quando è stato firmato il contratto di locazione, spende 471.000 euro di affitto. Il contratto scade nel 2021. Questi conti sono stati effettuati sulla base di documenti pubblici, difficilmente recuperabili grazie ad alchimie tra il barocco e il bizantino del nostro sito Internet, dal segretario dei radicali italiani Mario Staderini,

che, a fine contratto, ogni senatore, se mai ci entrerà, sarà comunque costato alle casse pubbliche una media di 8.000 euro al mese». Anche nel centro di Roma, credo che con 8.000 euro al mese si potrebbe far fronte ad un

La consegna del primo lotto era prevista nel 2006, poi slittata nel 2008, poi un'"aggiuntina" nel 2009 e adesso, nella relazione allegata all'ultimo documento del bilancio del Senato 2010, approvato un mese fa, si prevede finalmente «la consegna degli uffici entro l'anno». Ma con una postilla: occorre ancora una volta destinare significative risorse finanziarie all'acquisizione degli arredi, indispensabili alla funzionalità degli uffici e dei locali. Insomma, a spanne, manca ancora un milione per poter

Ci è stato detto, in risposta ad alcuni rilievi posti durante il dibattito generale generale sul bilancio del nostro Senato, che probabilmente l'edificio sarà pronto a fine legislatura. Sappiamo però che in Italia le legislature non hanno una scadenza fissa; quindi, in effetti, la concomitanza della fine dell'anno potrebbe sovrapporsi con la fine della legislatura. È chiaro che si tratta di decisioni pregresse, sulle quali la Presidenza credo possa tornare utilmente in questa sede, e magari con un comunicato ufficiale. che il modo in cui siamo chiamati a discutere del nostro bilancio interno non aiuta alla migliore gestione del denaro pubblico che ci viene affidato per poter svolgere nel migliore dei modi i nostri lavori.

che protestavano per la grave crisi che sta vivendo l'agricoltura sarda, in particolare il settore ovicaprino a causa del prezzo del latte. È da mesi che gli agricoltori sardi protestano. Ieri si sono verificati tafferugli tra le forze dell'ordine e i manifestanti, con lanci di lacrimogeni, il cui fumo ha invaso via Roma e le zone adiacenti il palazzo del Consiglio comunale. Il bilancio degli incidenti di ieri somiglia spaventosamente ad un bollettino di guerra:

che deve rimanere estranea alla protesta, riteniamo che ci sia stata una sorta di impreparazione a fronteggiare la pressione, assolutamente prevedibile, di gente che attende dal Governo impegni concreti per superare lo stato di crisi. Per tale motivo

a tutti i pastori che sono rimasti feriti, a tutti i cittadini che erano presenti che si sono trovati coinvolti e, se mi permettete, anche ai poliziotti che devono portare avanti il proprio lavoro e seguire delle indicazioni.Voglio ricordare che, oltre ai feriti

Chi mi ha preceduto ha già illustrato la situazione drammatica in cui versa l'industria agroalimentare in Sardegna.

un litro di latte oggi viene rimborsato meno di un litro d'acqua. È vero che è importante l'acqua nel nostro Paese, ma un litro di latte per essere prodotto richiede una fatica paurosa, nettamente superiore a quella necessaria per attingere acqua da un pozzo.

colleghi che facevano leva su battute spiritose o su barzellette, che rifiuto di fronte a tanta sofferenza. Io pretendo che anche i pastori della Sardegna ricevano attenzione come tutti i lavoratori d'Italia.

anche le considerazioni e la proposta appena rivolta alla Presidenza dalla senatrice Mongiello. Lo faccio come Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. tratta di un problema che tutti conosciamo, che si trascina effettivamente da parecchio tempo, che investe responsabilità in parte dei Governi nazionali e in parte di quelli regionali;

perché assume oramai una dimensione vasta, per risolvere le questioni che vi sono dietro, che - come è stato già detto - riguardano il prezzo del latte e la possibilità di far vivere la propria azienda e la propria famiglia. Per questi motivi ritengo

tutto quello che fa la politica, quello che fanno i palazzi del potere. Quindi, vengono messi giustamente sulla graticola per rendere conto del loro operato e della loro etica pubblica. *mass media*, giornalisti distratti, e non solo, fanno finta di non vedere, non hanno la stessa attenzione per ciò che avviene in alcuni santuari intoccabili del potere economico e di alcune autorità vigilanti.

per salvaguardare gli interessi delle banche. In questo atto di sindacato ispettivo mi soffermo sul fatto che - in data 21 luglio 2009 - è stato nominato commissario del Banco emiliano romagnolo un signore che si chiama Fernando de Flaviis. Ebbene, risulta che questo commissario, nominato dal governatore Draghi, è indagato per il reato di usura, come risulta dagli atti della procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno al numero 160305RG "Notizie di reato modello 21", relativamente al periodo in cui ricopriva la carica di direttore generale della Cassa di risparmio della Provincia di Teramo, Banca Tercas, tra il 1998 ed il 2005. Signor Presidente, non si può far finta di non vedere questi scandali che vengono coperti da parte non solo dei *mass media* ma anche di coloro che avrebbero il dovere di andare a vedere. Faccio queste cose tutti i giorni. Quindi, signor Presidente, ritengo che sia un compito della politica e dei rappresentanti eletti democraticamente porre tali questioni. Non è possibile che ci siano sepolcri imbiancati che non rispondono ad alcuno dei loro operati, e quando sollevo tali questioni, noto una certa

della politica, dobbiamo offrire trasparenza, comportamenti eticamente non riprovevoli, ma anche quelli che stanno lì, gli oligarchi, devono rispondere a qualcuno del loro operato. È una prassi che non rispondono mai a nessuno, neanche ai rappresentanti del popolo: una prassi che deve essere quanto meno accantonata e

come è giusto che ci sia da parte della Presidenza, come c'è stata, una sollecitazione al Governo per dare risposte a queste sue interrogazioni, come quella che ha richiamato, e che ci sia una risposta precisa per chiarire i termini delle considerazioni da lei svolte

prima di riprendere la discussione sul disegno di legge conosciuto come scudo costituzionale alle alte cariche dello Stato, i senatori del Partito Democratico chiederanno che il Governo, in quella sede o in altra, che è la Presidenza delle Commissioni senza essere costretti ad investire formalmente la Presidenza del Senato - venga convocato per riferire dei lavori della Commissione paritetica che redige le norme di attuazione sul nuovo regime delle entrate della Sardegna deciso dal Parlamento nazionale con la legge finanziaria adottata nel dicembre 2006. Questo era l'anno in cui il sistema doveva entrare a regime e consentire alla Regione di rispondere, tra l'altro, alle richieste di interventi strutturali e di emergenza nel settore agropastorale, la cui esplosione ha provocato ieri a Cagliari i fatti di cui questo ramo del Parlamento, pochi minuti fa, si è interessato e di cui dovrà tornare ad interessarsi con l'intervento in Aula del Ministro dell'interno e, come noi auspichiamo, anche del ministro dell'agricoltura Galan. A questa domanda di convocazione del Governo non c'è stata ancora una risposta. una risposta. È secondo noi lesivo di un'applicazione seria del principio di relazione leale e collaborativa che deve esistere tra lo Stato e la Regione il fatto che il Governo nazionale non abbia ancora chiuso chiuso una partita in cui l'esercizio 2010 - quello in cui devono entrare a regime le nuove regole - sta per finire e i denari non sono ancora arrivati, e la conseguenza è la strozzatura finanziaria di una Regione che non può più reagire minimamente alle urgenze sociali ed economiche che abbiamo davanti e che possono degradare, per le proteste che provocano, da problemi economici settoriali a problemi di ordine pubblico. Ritorneremo in Aula per sentire cosa diranno il Governo e la Presidenza della Commissione affari costituzionali su questa insistente richiesta del Partito Democratico.